In data 30 marzo 2007 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia:*

e mi espressi, in quell'occasione, sia utilizzando il condizionale e non l'indicativo, sia ipotizzando che si trattasse di un *gossip* giornalistico, ciò che lei stesso si augurò nel suo breve intervento di replica. Adesso, a distanza di due settimane, il settimanale «L'espresso» riporta una precisazione del senatore Russo Spena che si esplicita nei seguenti termini.

«è stato interpretato da un senatore di AN in maniera gravemente imprecisa». Rammento che l'articolo, che Russo Spena definisce «pur in sé preciso», diceva: «Dopo le ultime elezioni, Malabarba annunciò le sue dimissioni da senatore per lasciare il posto ad Haidi Giuliani. "Torno a fare l'operaio", disse, e a ottobre si dimise da Palazzo Madama. Non prima però di aver sottoscritto un vantaggioso accordo con il capogruppo di Rifondazione Comunista al Senato, Giovanni Russo Spena, per garantirsi un vitalizio senatoriale più ricco e il pagamento di un debito con l'INPS. Per tutta la durata della legislatura venivano infatti garantiti a Malabarba, a titolo di rimborso spese, 3.500 euro netti al mese, per 15 mensilità,

non mi può imputare pubblicamente di aver interpretato in maniera gravemente imprecisa. Io ho interpretato correttamente e ho usato il condizionale perché mi rifiutavo di credere che un senatore, con fondi pubblici, attraverso il Gruppo di competenza, avrebbe ricevuto delle somme come *bonus* per favorire l'abbandono di un seggio. Poiché il senatore Russo Spena mi ha detto qui, in quest'Aula, dopo il mio intervento, che in realtà la vicenda lui l'aveva sottoscritta ma non l'aveva capita molto bene, e che la somma ammontava solo a 120.000 euro

credo che a lei non sfuggano questi particolari e che quindi debba dare luogo ad una qualche consequenzialità attraverso una Commissione a tutela della mia onorabilità e di quanto accade in questo Parlamento.

8 febbraio 2007, n. 8, sul quale, con molta buona volontà e anche con molto buonsenso, avevamo raggiunto in Senato un accordo unanime, o quasi,

finanze dei Comuni l'onere delle modifiche strutturali per consentire l'entrata in vigore a pieno del decreto Pisanu.

(proprio perché, spendendo milioni di euro per due gambe di calciatori, potessero anche spendere qualche centinaio di migliaia di euro per le modifiche degli impianti), ci è stata rimandata indietro con un emendamento

indiscriminatamente agli oltraggi, violenze, resistenze a pubblico ufficiale l'aumento della pena base da tre a cinque anni perché sarebbe stato molto

commesse contro pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico. La Camera, con un emendamento che non credo sia frutto di una mente giuridica accorta,

L'articolo 583-*quater* è stato modificato in tal senso: «Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, in occasione di manifestazioni sportive,

che riguarda solo gli agenti in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. La dubbia costituzionalità di questo articolo è chiara a tutti: a tutti: non è possibile, almeno alla luce dell'articolo 3 della Costituzione, punire con pene diverse soggetti che commettono lo stesso fatto. fatto. Lo stesso fatto è commettere lesione contro pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico; la specificazione ulteriore che siamo di fronte ad una manifestazione sportiva non può modificare addirittura l'irrogazione della pena, spostandola da una più più mite ad una più grave. Segnalo queste due contraddizioni e, come relatore, sono in attesa del dibattito in Assemblea per capire se dobbiamo rinviare il decreto alla Camera con gli emendamenti presentati nelle Commissioni riunite o se, per la ragion di Stato, ci dobbiamo piegare e licenziare

e *tout court*, perché il provvedimento licenziato dal Senato aveva un suo fondamento di equilibrio ed è strano che la Camera abbia voluto modificarlo.

piuttosto significative, altre invece assai marginali. La prima osservazione che intendo fare, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, è quella che

anzitutto ricordare ai colleghi che abbiamo introdotto tale norma sostituendola alla previsione aggravata di resistenza a pubblico ufficiale, alla quale abbiamo ritenuto di dover apportare questa modifica interamente sostitutiva preferendo un reato di danno probabilmente si sarebbe consumato soltanto attraverso espressioni non dirette e comunque non di danno diretto nei confronti dei pubblici ufficiali, proprio per dare maggiore oggettività alla condotta. Qual è il paradosso che si è verificato, signor Presidente, e che vorrei illustrare, in aggiunta alle osservazioni del collega Di Lello Finuoli? La Camera ha ridotto la pena che il Senato aveva

segnatamente la pena da otto a sedici anni, è esattamente la pena oggi prevista per le lesioni gravissime in danno di pubblici ufficiali e, come potrei dire con un *coup de théâtre,* ve lo dimostro immediatamente.

la Camera dei deputati per le lesioni gravi è la reclusione da quattro a dieci anni. Signor Presidente, ci si è dimenticati che quando si tratta di lesioni gravi in danno di pubblici ufficiali scatta l'aggravante dell'articolo 61, n. 10, che aumenta di un terzo la pena. Quindi, oggi, a prescindere da questa norma, la pena per le lesioni gravi in danno di pubblici ufficiali è - non «sarebbe» - da quattro anni a

Analogamente, in caso di lesioni gravissime, la pena prevista dal codice penale è da sei a dodici anni. Se noi aumentiamo di un terzo, ai sensi dell'articolo 61, n. 10, la pena diventa da otto a sedici anni, che è esattamente quella prevista dalla Camera, con la sola differenza che la pena edittale che ho citato si applica in danno di qualsiasi pubblico ufficiale, in qualsiasi circostanza, in ragione della propria divisa;

e la sola differenza risiederebbe nel fatto che il Senato della Repubblica avrebbe introdotto un'ipotesi autonoma di reato, a differenza dell'ipotesi aggravata che è quella che ho citato. signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo così affidando al giudizio della Corte di cassazione, dei tribunali, la decisione se si tratta in realtà di un'ipotesi autonoma o di una circostanza aggravante e quindi stiamo affidando sostanzialmente ai magistrati e alla giurisprudenza la risoluzione di questo busillis che la Camera ha ritenuto di dover introdurre nel nostro ordinamento. Passo immediatamente all'articolo 10 per dire che anche in questo caso era assai preferibile la formulazione originaria del Governo. Voglio ricordare che allo stadio di San Siro per tre anni non sono state compiute quelle attività di sicurezza passiva previste dal decreto Pisanu che poi sono state realizzate, con scandalo giornalistico, in soli due giorni. Il Governo ci ha detto che ciò è accaduto non in ragione della cogenza di questo decreto, che tutti abbiamo apprezzato, ma della sanzione che avrebbe comportato il non consentire più delle partite la domenica. Credo che la cogenza di questo decreto, oggi e per il futuro, sia quella a cui dobbiamo fare riferimento, e allora signor Presidente, onorevoli colleghi, dire che le società possono provvedere a realizzare delle sicurezze passive senza oneri a carico della finanza pubblica sostanzialmente vuol dire che le società lo possono fare ma che gli enti non lo debbono pagare, in buona sostanza che non lo deve fare nessuno. nessuno. Anche qui, è di lapalissiana evidenza l'incongruenza che si è generata ed è stata opportunamente rilevata dalla Commissione. Altre questioni sono state rilevate dalla Commissione, come i biglietti gratuiti in favore dei minori infraquattordicenni, ottenibili dimostrando un legame di parentela entro il quarto grado che sfugge a ogni tipo di certificazione; avendo introdotto un regime nominativo dei biglietti, è difficile comprendere come si possa poi dimostrare questo legame di parentela, che non compare nemmeno sullo stato di famiglia. aspetto che va chiarito, e che riguarda invece le nostre dirette responsabilità, è che quando abbiamo previsto molto severamente e molto seriamente che il cosiddetto divieto di andare allo stadio dovesse essere applicato con sentenza immediatamente esecutiva era evidente che questa dovesse essere impugnabile attraverso i rimedi ordinari; è questa la ragione per cui sono stati ritirati quegli emendamenti che prevedevano delle impugnazioni speciali. Signor Presidente, ricordo qui le incongruenze che abbiamo rilevato, il lavoro della Commissione si è focalizzato essenzialmente su questi due punti e su un terzo che pure è affidato al lavoro emendativo e che risulta. Ovviamente, attendo di conoscere il parere dei Gruppi nell'Aula per formulare le mie considerazioni finali come relatore. Ci rendiamo perfettamente conto che i termini e i tempi

La ringrazio, signor Presidente, e in primo luogo mi consenta di ringraziare il Senato intero per il lavoro che è venuto svolgendo su questo decreto, migliorandolo in prima lettura e facendolo, per migliorandolo in prima lettura e facendolo, per di più, con un larghissimo consenso che è stato incoraggiante in presenza di un tema che ha coinvolto larghissimamente l'opinione pubblica e che ha suscitato sentimenti di reazione fortemente condivisi anche all'interno del mondo del calcio, saggiamente guidato, per nostra fortuna, in questi mesi dal commissario Pancalli, che proprio ora sta lasciando il suo incarico. È stato un bellissimo episodio parlamentare, anche se occasionato da una vicenda tragica,

con una rapidità che sembrava impossibile prima che tutto questo, ahimè tragicamente, accadesse. Ora siamo arrivati, nel gioco del nostro bicameralismo, alle battute finali, con un testo che il Senato si trova davanti e che non ritiene soddisfacente in alcuni punti particolarmente delicati. Ho ascoltato con grande attenzione le due relazioni e se dichiarassi di essere in disaccordo con quanto detto dai relatori direi francamente una bugia. Ho cercato di verificare nel codice penale, perché esistono fattispecie che configurano una maggiore gravità di trattamento per un dato comportamento in relazione a circostanze specifiche.

persona che ne è vittima. Trovo particolarmente arduo adottare una distinzione analoga nel caso di lesioni gravi o gravissime a danno di pubblico ufficiale, ancorché mi renda conto che il contesto sportivo crea particolari incentivi alla violenza e quindi induce a una particolare attenzione, ma sarebbe francamente arbitrario concludere che non vi siano altri contesti nei quali vi è una situazione analoga, per cui potrebbe essere difficile da parte della Corte costituzionale ritenere ragionevole tale differenziazione nella gravità.

e percepisco che modificarlo ora lo mette a rischio.

decreto. Possiamo aggiustarlo dopo (anche immediatamente dopo), ma non ci assumiamo la responsabilità del rischio grave che possa non essere approvato questa settimana

di far approvare dal Governo, tra oggi e domani, un secondo decreto‑legge che corregga il primo. Non siamo in condizioni di farlo, perché si corregge dopo essersi accorti di aver commesso un errore: non si può chiedere al Capo dello Stato di firmare contestualmente la legge di conversione che già abbiamo detto essere sbagliata e l'atto che la corregge. Al Capo dello Stato dobbiamo riservare il ruolo di garante della nostra correttezza, non di garante dei difetti della nostra incapacità di coordinarci a dovere e di rispettare i termini costituzionali. Non ci sentiamo di chiedere al Capo dello Stato di assolvere questa parte. però, prontissimi a sostenere una iniziativa legislativa, anche immediata, che venga dal Senato, nelle forme, nei modi e nei termini che i Capigruppo vorranno determinare, determinare, affinché si provveda immediatamente dopo. Il vizio di questa legge di conversione ha un suo ha un suo peso, ma rischiare di far cadere l'intero decreto in ragione di tale vizio comporta un costo che, francamente, supera il beneficio che possiamo ottenere immediatamente dopo. vi chiedo - lo chiedo a tutti -, consapevole delle ragioni contrarie che militano nei confronti della mia richiesta, di votare la legge di conversione, il testo che per taluni aspetti non vi piace arrivato dall'altra Camera. Si provvederà subito a rimediare, ma intanto mettiamo al sicuro ciò che è importante mettere al sicuro. Vi ringrazio per quello che vorrete fare.

vorrei subito chiarire al ministro Amato, con il quale abbiamo avuto modo di interloquire anche fuori dal dibattito, che il Gruppo di Alleanza Nazionale non vuole assolutamente atto un'operazione ostruzionistica per far cadere il decreto. Prendo la parola proprio per sgomberare il campo da questo dubbio. Tuttavia, signor Presidente, faccio appello a lei: possiamo approvare questo decreto con le modifiche dei due emendamenti,

Non abbiamo svolto un'azione ostruzionistica per rispetto a lei, signor Presidente, perché lei, prima che in Conferenza dei Capigruppo sollevassimo il problema, ci ha comunicato di aver scritto al presidente della Camera Bertinotti, facendo notare l'anomalia. l'anomalia. Non possiamo farci carico tutte le volte di rimediare ai problemi della Camera. Ora siamo di fronte ad un decreto che tutti vogliamo convertire (o comunque

responsabili dei Gruppi dell'opposizione, per cercare di trovare un'intesa e mi pare che gli abbiamo dato la massima collaborazione. Ma è evidente che il Capo dello Stato non può

i colleghi - e noi assicuriamo la massima collaborazione - a far sì che il provvedimento sia approvato prima della fine della seduta di questa mattina, in modo che torni

che questi emendamenti siano approvati; allora ce lo dica, perché il problema diventerebbe politico e anche il nostro atteggiamento sarebbe diverso. Se c'è qualcuno che mette i bastoni fra le ruote non è l'opposizione:

Presidente, le Commissioni riunite 1a e 2a hanno lavorato, anche in occasione della seconda lettura, in modo particolarmente efficace, registrando tra l'altro un consenso unanime.

riguardo all'eccezionalità dell'evento «violenza negli stadi» e all'opportunità che il decreto venisse convertito in tempo, di ridurre soltanto a due

per l'atteggiamento non solo collaborativo, ma devo dire di vivo interesse con cui hanno contribuito alla qualità dei nostri lavori. È

Il Regolamento più lasco della Camera, da un certo punto di vista più garantista per le opposizioni per quanto riguarda la discussione dei decreti-legge, rischia però di trasformarsi ogni volta in un capestro per il Senato.

e credo della assoluta necessità - di convertire un decreto-legge, lo dico probabilmente con un particolare*pathos*, che è stato voluto dal Governo con grande tempestività, dopo i fatti di Catania e dopo l'uccisione dell'ispettore Raciti. Ora, penso che sarebbe assolutamente incomprensibile per qualunque cittadino italiano assistere al paradosso di un disegno di legge di conversione, approvato all'unanimità in ciascuna delle Camere, che però non riesce a convertire per tempo il decreto.

di concordare tra i Capigruppo di maggioranza e di opposizione un disegno di legge che valga ad introdurre nell'ordinamento le modifiche volute dalle Commissioni in questo ramo del Parlamento. Credo che tale soluzione

dare a quest'Aula la possibilità di convertire il decreto con modifiche condivise dall'unanimità delle Commissioni entro la fase antimeridiana della giornata.

Signor Presidente, qui è in gioco il sistema del funzionamento bicamerale, non ne faccio una questione campanilistica: sono contento di non farla, proprio su un tema condiviso - negli emendamenti che oggi ci troviamo a discutere - da parte di maggioranza e opposizione.

Ci troviamo dinanzi una correzione condivisa dallo stesso Governo, e senza nessuna vena di polemica, mi creda, signor Ministro, lei conosce la stima che ho nei suoi confronti mi chiedo come mai l'Esecutivo non sia riuscito a fare in modo che il percorso della Camera su questo testo che oggi non è condiviso potesse essere contrastato con i normali mezzi parlamentari che ci riconosce la Costituzione; oggi non ci troveremmo qui a dover discutere ulteriormente. Ci troviamo dinanzi a un'esigenza condivisa di carattere quasi costituzionale: dico «quasi» perché, a mio avviso, siamo ai limiti della Costituzione, ma siamo, sicuramente, nel baratro dell'inaccettabilità sostanziale, perché vi sono proposizioni che cozzano diametralmente contro i principi del nostro impianto giuridico. Un reato è un reato a prescindere dal luogo in cui viene posto in essere;

perché quando si paventa il pericolo della decadenza - e lo si fa da parte dei vertici della Camera dei deputati - credo che in sostanza Sostanzialmente si dice al Senato di non esercitare la sua funzione legislativa,

- ciò accadrebbe in quanto la Camera entro gli otto giorni che avrebbe per poterlo convertire non si sarebbe dotata dei tempi e delle possibilità per approvarlo definitivamente, ma la responsabilità non sarebbe certo di questo ramo del Parlamento, che avrebbe esercitato la sua corretta funzione.

di essere un'opposizione responsabile e proprio titolari e reduci di quell'atteggiamento ci sentiamo oggi legittimati a rivolgere un appello alla maggioranza e al Governo

insistiamo su questa possibilità. Non ne facciamo una questione di principio, ma una questione di corretto e reciproco rispetto del funzionamento della Camera e del Senato. Esiste una Costituzione, esiste un bicameralismo: esercitiamo il nostro ruolo consapevoli del fatto che stiamo chiedendo

abbastanza paradossale che si arrivi in Aula in questa situazione. Credo, infatti, che questa discussione sarebbe dovuta avvenire utilmente in Commissione. Ritengo che le legittime per certi versi condivisibili - argomentazioni del Ministro sarebbero state molto più utili in quella sede; peraltro, non ci avrebbero messo nella situazione

Un'ultima considerazione che mi induce ad essere contrario ad un provvedimento di sospensione, sia pure breve,

era stata data la disponibilità da parte dello stesso Esecutivo ad emendare, anzi ad abrogare con successivo provvedimento d'urgenza e non ordinario, questa norma della quale si sta discutendo.

la profonda consapevolezza e la convinzione da parte di tutti i Gruppi del Senato che gli emendamenti approvati dalle Commissioni sono assolutamente utili e necessari. chiesto congiuntamente di ascoltare una comunicazione del Governo, che sarà fatta in Aula, circa le modalità con cui si possono raggiungere gli obiettivi che il Senato chiede. Sulla base di questa valutazione, i Gruppi i Gruppi sono disponibili a proseguire l'esame in modo tale da non far decadere il decreto.

ritiene che la strada migliore sia quella di una iniziativa legislativa, che nasca all'unanimità all'interno del Senato, e che può essere - ritengo - varata se ci sono i consensi (e ci sono) in Commissione in sede deliberante al più presto: essa avrà il sostegno del Governo

dove il ministro Chiti ha già operato le prime verifiche che lo portano a ritenere che l'urgenza sarà comunque votata affinché abbia corso e dove riteniamo che il provvedimento correttivo avrà corso nei termini che i senatori riterranno di definire. Questa Questa strada è preferibile rispetto ad altre, perché si muove sul duplice terreno dell'errore politico e della possibile incostituzionalità delle norme diverse approvate dalla Camera e se nel cambiamento giocano insieme un motivo di orientamento, di *policy*, di valutazione politica, e uno di possibile incostituzionalità, ciò è molto meglio anche ai fini della conduzione alla promulgazione della legge di conversione, in merito alla quale vi rinnovo la richiesta che sia approvata nel testo, non interamente gradito, ricevuto dalla Camera.

ci siamo riuniti e abbiamo ascoltato con interesse quanto detto dal Ministro, che va nel senso delle intese raggiunte in maniera informale durante la pausa dei nostri lavori. A noi sta a cuore, signor Presidente, che questa novella legislativa che ci accingiamo ad attivare tra poco, terminata la conversione del decreto, credo senza modifiche, non soltanto possa essere approvata al più presto dal Senato ma abbia il sostegno del Governo, come ha detto il Ministro; infatti, secondo noi, signor Presidente (l'ho detto poc'anzi nella riunione), è più un problema del Governo che non dell'opposizione andare a spiegare dopodomani alle forze dell'ordine

senza precedenti e credo possa costituire un messaggio negativo nei confronti di chi, rischiando la vita, si occupa della sicurezza del nostro Paese. ci siamo fatti carico di sollevare questo problema con gli emendamenti, che avevano trovato il consenso della maggioranza, proponendo una modifica di buonsenso. Ci siamo fatti carico anche dell'esigenza di evitare di dare alibi a qualcuno perché il decreto possa non essere convertito, perché ci sta a cuore mostrare al Paese, a tutti i cittadini e alle stesse forze dell'ordine che il Parlamento è intervenuto unanimemente per dare un segnale forte e chiaro. Naturalmente auspichiamo che questo percorso legislativo possa essere più agevole, e non solo in Senato, dove saremo noi a gestirlo e non ho motivo di avere preoccupazioni in tal senso.

voteremo questo testo, non condividendone alcune parti, nell'interesse superiore della collettività, ma è evidente che spiegheremo al Paese e alle forze dell'ordine che l'entrata in vigore di tale provvedimento, che contiene una norma riguarda le sanzioni di un reato che tocca proprio chi lavora per la sicurezza del Paese, non è responsabilità dell'opposizione ma di un Governo e di una maggioranza, che comunque si sono fatti carico di intervenire al più presto. A ognuno il proprio ruolo,

tocca la sensibilità e la coscienza di chi rischia la vita per salvare i nostri cittadini e di chi serenamente ha il diritto-dovere di vivere in pace nel nostro Paese. Lo facciamo perché ci sta a cuore questo,

Presidente, questa decisione non ci piace, la subiamo perché non vogliamo assolutamente correre il rischio che il decreto non sia convertito. Chiedo, però, che oggi stesso sia scritto il testo del disegno di legge, che sia firmato dai Capigruppo nelle Commissioni di competenza, che domani sia discusso e possibilmente approvato in Commissione e la prossima settimana si possa chiedere la sede deliberante. Credo che almeno questo si debba fare. Naturalmente, se c'è il consenso dell'Assemblea del Senato, gradirei anche, però, che da parte del Governo ci fosse una parola di condivisione di questo percorso. Soltanto in tal modo potremo accettare questo accordo, questa mediazione che ci costa molto, perché approvare un provvedimento in cui è chiaro che ci sono profili di incostituzionalità non piace a nessuno, ma l'emergenza e la situazione sono tali e nel Paese questo

colleghi, d'intesa con il presidente Bianco, abbiamo convenuto di convocare al più presto, anche nella giornata di domani, le Commissioni riunite;

della parte largamente prevalente delle Commissioni, ritiriamo i tre emendamenti presentati. Mi consenta, con l'occasione, di fare delle considerazioni molto rapide. La prima, signor Presidente, è che esiste un'asimmetria istituzionale tra Camera e Senato che va prevede, nell'esame dei decreti-legge, la regola della ghigliottina entro il trentesimo giorno, che comporta il contingentamento dei tempi, la decadenza degli emendamenti, la necessità di voto finale. La Camera non solo non ha una normativa di questo tipo, ma ha ritenuto anche di applicare la normativa nel senso del divieto del contingentamento dei tempi nella decretazione d'urgenza. Si potrà, in futuro, riformare il bicameralismo, ma finché permane il sistema del bicameralismo perfetto e paritario non è non è accettabile che ci sia questa asimmetria istituzionale. La prego pertanto di valutare le iniziative opportune per evitare che questo si ripeta. Le altre due rapide considerazioni sono di merito. Le Commissioni riunite, pur avendo dubbi e perplessità, come è normale, su altri aspetti delle modifiche apportate dalla Camera, non hanno avviato questo confronto per un ripicco, come si legge anche sui quotidiani. Ci sono due norme che saranno oggetto del disegno di legge di cui si sta parlando, la prima delle quali è incostituzionale, come il ministro Amato ha confermato questa mattina, per di più potendo farlo dall'alto della sua dottrina che tutti gli riconosciamo. La seconda, di cui si parla meno, nasce da un intervento della stessa *lobby* che dopo la morte del povero ispettore ebbe a dire che i morti fanno parte del sistema e che ha fatto pressioni per evitare che fosse posta a carico delle grandi società sportive, che del circuito calcistico hanno tutti i vantaggi e vorrebbero averne senza pagarne i costi, con l'esonero dalle spese per le ristrutturazioni degli stadi. Si è aggiunto inoltre, per venire incontro alle giuste richieste dell'ANCI, che non sono nemmeno a carico dei Comuni; rimane il fatto che stiamo varando una legge in cui si dice che gli stadi devono essere ristrutturati per ragioni di sicurezza ma che nessuno è tenuto a pagarne le spese. Non è giusto, però, che a pagarle sia Pantalone, ma è giusto, in una logica di mercato della quale tanto si parla, che i costi economici siano a carico di coloro che ne ricavano ingenti benefici economici. Questa seconda, altrettanto rilevante della prima, è la ragione per la quale le Commissioni riunite avevano approvato concordemente quei due emendamenti. A me fa piacere che quel clima di concordia si sia mantenuto questa mattina nella riunione con il Governo, da parte delle Commissioni 1a e 2a del Senato, fra maggioranza e opposizione; in questo modo,

Signor Presidente, non vorrei rovinare il clima di concordia e di «volemose bene» che si è instaurato in questo momento, ma devo dire che, se prima avevamo delle forti perplessità, la riunione testé conclusasi ce le ha rafforzate. Sotto un certo punto di vista devo anche fare i complimenti al Governo, perché dopo una serie di errori molto gravi che ha fatto nella conduzione del provvedimento riesce, con un doppio salto mortale carpiato rovesciato, a ribaltare la situazione nella direzione auspicata. Peccato che ci sia una vittima: è il Senato, che esce profondamente umiliato dalla vicenda. dalla vicenda. Quali sono stati gli errori del Governo? Primo: non è stato capace di coordinare i Gruppi della maggioranza, perché è evidente che su un decreto-legge la maggioranza ha

(dove avrebbe dovuto essere innescata, cioè in Commissione), ma lascia che il problema si trascini fino all'ultimo minuto: arriva in Aula, ci pone di fronte al fatto compiuto

i signori deputati hanno nove giorni, ma sostengono di non poter convertire il provvedimento. Non possono convertirlo perché non vogliono, signor Ministro; lei lo sa benissimo, perché dalla Camera ci hanno già fatto sapere (se lo hanno fatto sapere a noi, sicuramente lo hanno fatto sapere anche a lei) che il Senato non deve osare toccare quelle norme,

di poter votare un testo che non soltanto è anticostituzionale, ma contiene una norma - mi riservo di ritornarci in sede di dichiarazione di voto - veramente scandalosa, che è una vittoria della sinistra oltranzista, una delle tante che dobbiamo subire in questa legislatura.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei spendere appena due parole. Voglio dire innanzitutto che mi pare non ci sia equivoco tra di noi.

in realtà prevede una sanzione che sarebbe comunque raggiungibile a codice vigente, bastando l'applicazione delle norme che prevedono l'aggravante ordinaria del fatto commesso nei confronti di pubblico ufficiale

più grave la previsione che sposta dal dovere alla facoltà ciò che originariamente avevamo previsto come un obbligo per le società sportive di adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza. Non trascurerei anche l'ulteriore emendamento, quello che richiede che il pericolo sia concreto, perché non sfugge a nessuno come questa norma - proposta tra l'altro dall'onorevole Pecorella e non dalla sinistra radicale - necessariamente attenua il il vigore della previsione anche sanzionatoria. Credo che oggi non stiamo commettendo un atto di lesa maestà nei confronti del Senato. Stiamo al contrario - grazie alla disponibilità, all'intelligenza e alla responsabilità anche dei colleghi dell'opposizione, in particolare dei colleghi Schifani, Matteoli e D'Onofrio - celebrando la responsabilità di questo ramo del Parlamento di fronte a una questione così complessa, delicata e simbolicamente significativa. Credo che le vittime in tutta questa vicenda siano soltanto i rappresentanti delle forze dell'ordine, che pagano con la vita come nel caso dell'ispettore Raciti - e tutti quei cittadini che vogliono godere tranquillamente una bella domenica e una bella giornata di sport e che, in ragione delle violenze operate durante le manifestazioni sportive, vedono sacrificato questo diritto proprio e delle proprie famiglie. dunque, la posizione del nostro Gruppo e confermo, per quanto riguarda il Gruppo dell'Ulivo, la piena, assoluta disponibilità non solo, ovviamente, alla presentazione immediata del disegno di legge, come dicevano i colleghi Bianco e Salvi, ma anche alla sua più rapida approvazione, in questo e nell'altro ramo del Parlamento.